L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE i senatori Luigi Augussori, Gianluca Castaldi, Gianluca Ferrara, Renato Schifani, Paola Taverna, Achille Totaro e Vito Vattuone. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima delegazione i deputati Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE i senatori Luigi Cesaro, Giovanbattista Fazzolari, Patty L'Abbate. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima delegazione i deputati Stefania Ascari, Marco Maggioni, Raphael Raduzzi, Debora Serracchiani. Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo il senatore Giuseppe Moles. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima delegazione i deputati Giulio Centemero e Yana Chiara

Commissione, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

la notizia della morte di bambini dimenticati in auto desta sempre sconcerto e incredulità nell'opinione pubblica, ma purtroppo non rappresenta una novità. In quest'Aula non possiamo rimanere indifferenti di fronte a casi drammatici come quelli che abbiamo conosciuto e dobbiamo attivarci a tutela di questi innocenti, ma anche dei loro genitori e dei loro cari, evidentemente stressati dai ritmi incalzanti di una società, quella odierna, che logora la vita quotidiana e vittime di un meccanismo di *blackout* inspiegabile nella memoria. Le motivazioni sono di solito la fretta, lo *stress* e l'affaticamento mentale, che affliggono gli adulti di ogni genere ed estrazione sociale nelle società contemporanee, per cui i bimbi vengono dimenticati perché si pensa di averli lasciati a scuola, dai nonni oppure a casa. La tecnologia ci permette ormai di ovviare a questi crudeli scherzi della psiche, offrendo soluzioni in grado di prevenire e ovviare ai pericoli derivanti dai ritmi intensi della vita quotidiana. L'Italia, già in prima linea in materia di sicurezza stradale, nel momento in cui il provvedimento che stiamo esaminando sarà approvato sarà all'avanguardia anche per la tutela della vita dei nostri figli. Questo provvedimento dà infatti attenzione ai più piccoli ed è volto a scongiurare i tanti casi di morti assurde. Solo per fare l'esempio degli Stati Uniti, qui muore nell'abitacolo dell'auto di famiglia un bambino ogni dieci giorni, con una media di 37 vittime l'anno. Sono dati agghiaccianti, che devono imporre una riflessione. Negli ultimi anni troppi i tragici eventi che, anche in Italia, hanno riempito le cronache e sconvolto l'opinione pubblica. Dal 2011 ad oggi si sono verificate ben sette tragedie, troppe, che vanno sicuramente evitate. La proposta di legge che oggi discutiamo in quest'Aula vuole parlare alle famiglie, dare risposte, partire da quelle tragedie affinché non ve ne siano altre. A tal fine, l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, prevedendo che, quando si trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni, assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, si ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme, rispondente a determinate specifiche tecniche, volto a prevenire l'abbandono del bambino. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme

approda oggi in Aula il testo approvato dall'8a Commissione, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Desidero innanzi tutto ringraziare i colleghi di tutti i Gruppi per il lavoro svolto in 8a Commissione che ha portato ad una rapida approvazione di un testo la cui finalità è ampiamente condivisa. Il disegno di legge è stato infatti approvato dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 20 settembre 2018. Questo provvedimento è, ai fini della sicurezza dei bambini più piccoli, un passo assolutamente importante, invocato da tempo per tutelarli dal rischio di essere inconsapevolmente dimenticati nell'abitacolo delle autovetture chiuse, veicoli che, come ricordava il collega Ruspandini, possono diventare delle vere e proprie trappole mortali. Ricordo che secondo i dati presentati dal produttore del primo dispositivo antiabbandono, in audizione in Commissione trasporti alla Camera, nel 2008 ci sono stati già 45 casi. Nel 2014 un genitore su quattro ha ammesso che gli è successo almeno una volta di dimenticare il figlio in auto e solo fortunatamente non si è arrivati alla tragedia. Passando all'*iter* e all'esame del testo, la Commissione ha esaminato, in sede redigente, il disegno di legge n. 766, congiuntamente a diversi disegni di legge presentati da altri Gruppi. La proposta di legge n. 766, già approvata dalla Camera dei deputati, è stata adottata come testo base e approvata nell'identico testo trasmesso dalla Commissione trasporti della Camera. La Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni informali. In particolare, abbiamo ascoltato le imprese produttrici che hanno evidenziato la necessità di definire in sede ministeriale alcuni aspetti di natura tecnica relativi, ad esempio, all'omologazione dei dispositivi. Hanno inoltre avanzato la possibilità che siano le case produttrici automobilistiche a provvedere direttamente a dotare i veicoli di sensori di allarme. Sono stati presentati una decina di emendamenti al testo. Alcuni di questi sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno poi accolti dal Governo. Voglio in questa sede soffermarmi in particolare sul tema posto nell'ordine del giorno a prima firma del senatore Mallegni, che merita sicuramente un approfondimento futuro da parte della Commissione, ossia quello che gli autobus siano obbligatoriamente provvisti del sistema di ritenuta di tipo omologato. *(Brusio)*. il tono della voce nei discorsi tra di voi. DESSI' *(M5S)*. Nel merito, il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, introducendo un nuovo comma, 1-*bis*, che prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 ed N3 autovetture, gli autobus e i pullman fino a nove posti, e tutti gli autocarri fino alla massima portata, immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residente in Italia quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecniche costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, si introduce tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopraindicato. La violazione dell'obbligo è punita quindi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro. In caso di recidiva nell'arco di un biennio, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici Sempre all'articolo 1, comma 2, si prevede che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si prevede, infine, al comma 3, che l'obbligo di installazione del dispositivo d'allarme, si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere, in ogni caso, dal 1° luglio 2019. L'articolo 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. Gli oneri per la realizzazione delle campagne informative sono quantificati in 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme e prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, dispone che con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. A tale ultimo riguardo, sappiamo che sul reperimento delle risorse per le agevolazioni vi è un preciso impegno del nostro ministro Toninelli. Concludo la mia relazione ricordando che l'approvazione del provvedimento in esame è solo un primo passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che tutti abbiamo condiviso, cioè quello di garantire la sicurezza ai nostri piccoli e ai soggetti più deboli in ogni caso. *(Applausi dai

potrà sicuramente evitare tante tragedie. L'obiettivo del Governo e della maggioranza parlamentare è infatti quello di puntare a diminuire le vittime di sulle strade italiane, dove ormai contiamo una media di circa 3.500 vittime all'anno, ma sicuramente anche quello di puntare a una diminuzione di questo tipo di morti, che può essere facilmente evitato, anche grazie alle nuove tecnologie.

deputati. Intervengo in dichiarazione di voto sull'articolo 1, che, come veniva ricordato dai relatori, introduce dispositivi di allarme obbligatori per evitare l'abbandono dei bambini. di un tema rilevante, perché alla morte di un figlio si va ad aggiungere l'angoscia del senso di colpa, per un momento di amnesia, di dimenticanza, che poi una persona si porta dietro per tutta la vita e che acuisce ancora di più il dolore già grave per la perdita di un figlio. Non sta evidentemente a noi capire quali possano essere le cause che fanno arrivare a questo; tuttavia, quando i casi sono ripetuti, come è successo negli ultimi tempi, è importante prevenire e trovare dei sistemi affinché questi casi non si verifichino nuovamente. Da ciò deriva l'idea di modificare il codice della strada e di introdurre delle sanzioni amministrative, esattamente come per le cinture di sicurezza e per il seggiolino,

elemento introduce un obbligo e dispone delle sanzioni, come è importante che sia. La definizione delle caratteristiche del dispositivo sarà rinviata a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che deve essere emanato entro sessanta giorni; l'obbligo dell'installazione di questo dispositivo scatterà dopo centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. È importante che il decreto sia approvato nei termini

Signor Presidente, Elena due anni, Jacopo undici mesi, Giorgia un anno, Luca due anni. Questi sono i nomi di alcuni bambini che hanno perso la vita in Italia negli ultimi anni perché dimenticati in auto.

possono provocare dei vuoti di memoria anche a chi magari in passato, ascoltando queste notizie, asseriva che non gli sarebbe mai capitato. Può invece capitare a tutti. I fatti di cronaca riportano di tragedie analoghe sempre più frequenti anche all'estero; si tratta di un fenomeno che, seppur marginale (si parla di uno o due casi all'anno), non va trascurato. Queste tragedie vanno evitate a tutti i costi. la tecnologia ci consente di installare dei dispositivi che avvisano l'adulto quando chiude l'auto al cui interno c'è ancora un piccolo ospite. Il ministro Toninelli, sin dal primo suo insediamento, ha promesso di porre termine a questa piaga dell'abbandono e il MoVimento 5 Stelle si è dimostrato sempre molto sensibile a questo argomento ed ha voluto fortemente supportarlo a livello legislativo, votando a favore di un disegno di legge che impone l'obbligatorietà di questi dispositivi antiabbandono e che ha messo d'accordo anche le altre forze politiche. Pensare anche ad un solo bambino che muore in queste circostanze è qualcosa che tocca la sensibilità di tutti. Il disegno di legge andrà ad integrare l'articolo 172 del codice della strada, che regola l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. I più importanti fabbricanti italiani di prodotti per l'infanzia, che hanno partecipato alle audizioni preparatorie del disegno di legge, come diceva prima il relatore, stanno già tracciando la strada per la produzione di questi dispositivi, anche in considerazione delle entrate in vigore dell'obbligatorietà nel 2019. È importantissimo, infine, ricordare che prima ancora dell'obbligatorietà dei dispositivi antiabbandono, c'è quella dei dispositivi per la sicurezza dei bambini in auto. Secondo l'ISTAT, nel solo 2017 nel nostro Paese sono morti ben 25 minori di quattordici anni in incidenti stradali, e più di 8.000 sono rimasti feriti.

del Governo, onorevoli colleghi, nessun amore è più grande, nella vita di una persona, di quello che si prova per un figlio. E un solo dolore è ancora più intollerabile, per un genitore che perde un figlio: essere responsabile della sua morte. Non sono mai riuscita, neanche lontanamente, a immaginare cosa abbiano potuto provare quei poveri genitori colpiti da *blackout* al momento della presa di coscienza; ho pensato solo che con la morte di quel bambino finiva la vita di un'intera famiglia e anche, a volte, di una comunità. Non si può pensare che un'azione del genere possa mai essere compiuta per mera leggerezza, ma sicuramente è dovuta a un insieme di concause derivanti probabilmente dallo *stress* quotidiano. Perché tragedie del genere non si ripetano, Forza Italia ha presentato anche in Senato un disegno di legge, a cui se ne sono aggiunti altri delle diverse forze politiche, per rispondere a una questione sociale, purtroppo, meno rara di quanto si pensi e che, come ha ricordato la collega Bini, prima firmataria, come me, di un disegno di legge, non può che unire il Parlamento in un'unica voce. Avremmo voluto perfezionare ulteriormente il provvedimento, alla luce degli approfondimenti della discussione in Commissione e delle audizioni effettuate, ma, per riuscire a rendere operativa la legge entro l'estate, che è il momento dell'anno più a rischio, è necessario approvarla al più presto. L'articolo 1 del disegno di legge apporta proprio le modifiche all'articolo 172 del codice della strada rendendo obbligatoria l'installazione di dispositivi antiabbandono. Siamo comunque perfettamente consapevoli che quando si impone l'obbligatorietà di un sistema si altera un equilibrio, quindi siamo a maggior ragione consapevoli che ci ritroviamo a legiferare introducendo una regola etica che rischia di pesare economicamente su chi dovrà rispettarla, cioè i cittadini genitori. Per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti, che abbiamo trasformato in ordini del giorno perentori, sul cui recepimento da parte del Governo vigileremo, e che vanno dai minori oneri per i genitori al prolungamento del tempo di entrata in vigore della legge dei sistemi. Confidiamo che mai più tragedie del genere dovranno avvenire, perché un solo bambino salvato avrà dato un senso a questa legge.

in quest'Aula forse si parla troppo poco dei nostri figli, specialmente dei bambini nei loro primi anni di vita, anni in cui sono più vulnerabili, in cui è affidato ai genitori il compito di proteggerli e salvaguardarli contro ogni tipo di pericolo. Ma siamo esseri umani e anche il genitore più amorevole può sbagliare ed allora è lì che lo Stato, in questo caso il Parlamento, deve prevedere norme per difendere i più deboli. La vita che conduciamo tutti i giorni troppo spesso è carica di pressioni e di stress che si ripercuotono sulla nostra attenzione. Se parliamo di veicoli stiamo assistendo alla proliferazione di dispositivi tecnologici atti ad intervenire in caso di disattenzione: si chiamano ADAS (sistemi avanzati di assistenza per la guida) e il Parlamento europeo ha già approvato la proposta di renderli obbligatori per tutte le auto di futura costruzione. Si deve stabilire ancora da quando scatterà l'obbligo, ma sembra che a partire dal 2021 questo diventerà effettivo. Ma cosa è stato fatto per salvaguardare i bambini che viaggiano a bordo delle nostre automobili? L'impostazione che ha dato il Parlamento europeo con gli ADAS è un segnale importante, ma nulla è stato fatto per introdurre dispositivi di allarme per rilevare la presenza di bambini in auto, obbligando i produttori di seggiolini ad implementarli sui nuovi prodotti questo non può che essere fatto in sede europea. È per questo motivo che il Parlamento italiano si è fatto promotore di una norma diversa, che fa da apripista per tutto il nostro Continente. Con questo testo si introduce l'obbligo, per chi trasporta minori fino ai quattro anni di età di dotarsi di un dispositivo di allarme che finalmente azzeri il triste dato dei bambini morti perché abbandonati all'interno di un veicolo. Voglio ricordare come siano almeno nove i bambini che in Italia, dal 1998 ad oggi, hanno perso la vita per questa causa. Solo quest'anno, secondo i dati presentati dal produttore di dispositivi antiabbandono Remmy, ci sono già state 45 segnalazioni di genitori che hanno dimenticato i figli in auto, senza contare tutti quelli che non sono stati denunciati perché ovviamente in un genitore che ha una tale dimenticanza prevale un sentimento di vergogna che lo spinge a coprire ciò che è accaduto. Non siamo qui per accusare nessuno di alcuna cosa, anzi se come già detto porteremo a zero il numero delle morti per questa causa sarà un esempio di civiltà che il nostro Paese darà a tutti. Il testo di questa legge ovviamente rimanda al Ministero l'identificazione delle specifiche tecniche che questi dispositivi dovranno avere e in particolare di capire quali sono, tra i dispositivi presenti sul mercato, quelli più sicuri per i nostri figli. Non solo, il Governo ha già confermato come l'intenzione sia quella di salvaguardare questa norma - una iniziativa senza dubbio trasversale e di buon senso - da qualsivoglia speculazione. Il costo di questi dispositivi non deve ricadere sulle famiglie italiane: per questo è in valutazione l'inserimento, nella legge di stabilità, di un fondo per le detrazioni per il loro acquisto. Auspico che ci sia unanimità nel votare favorevolmente questo provvedimento e che in futuro le opposizioni possano convergere più spesso con la maggioranza su temi di fondamentale interesse generale, senza trincerarsi su posizioni precostituite.

discutere e prendere la parola su un provvedimento che chiama in causa sentimenti ed emotività. Come è stato già ricordato, infatti, questo provvedimento è una reazione ed una risposta a delle sciagure

di Pisa, e non è l'unico episodio. Si parla in questi casi giornalisticamente di drammatiche fatalità; si parla di un eccesso paradossale e incomprensibile di distrazione dell'effetto devastante di condizioni di stress emotivo e psicofisico. Non sta a noi giudicare. Si parla tecnicamente

2 prevede, infatti, che sia fornita un'informazione adeguata sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo 1, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. È anche prevista la copertura finanziaria dei relativi oneri. La disposizione specifica, infine, che i messaggi delle campagne costituiscono messaggi di utilità sociale; anche questo è un valore aggiunto del

politica, rispetto alla sua vocazione principale, ha allora la grande occasione di fare una cosa concreta che può salvare una e più vite. Il collega Ruspandini ha ricordato a quest'Aula i sette casi di bambini che sono scomparsi. Non voglio inchiodare la vostra emotività, ma questi casi non ci sarebbero stati se ci si fosse stata in questo Paese una legge apposita

l'obbligo per tutti gli autoveicoli su cui viaggiano i bambini di installare dispositivi dotati di un segnale sonoro e/o luminoso che allerti il conducente di una situazione di rischio e di pericolo, nel caso in cui i bambini restino all'interno del veicolo. È la risposta alla terribile espressione «amnesia dissociativa», quel *blackout* della memoria che nessuno può spiegare,

accorato, che è stato raccolto da tutti e questo - ripeto - è un bel segnale dato dalla politica. È un segnale perché i tempi sono stati rapidi, sia alla Camera che al Senato - agosto e poi settembre nelle Commissioni competenti

abbiamo la possibilità, in comunità di intenti, di dare a questo Paese una misura per salvare delle vite umane e, se anche ci fosse un caso soltanto sono molti di più, stando alle cronache), non solo avremmo svolto il nostro dovere, quello che ci porta qui a rappresentare i cittadini, ma avremmo assicurato un servizio al Paese, ai bambini e ai genitori. Non è allora un appello fatto soltanto al cuore, ma alla nostra responsabilità

un argomento delicato e sentito. Già nella scorsa legislatura il mio Gruppo aveva presentato alla Camera un disegno di legge a questo proposito, come in questa legislatura la senatrice Gallone è la prima firmataria di un disegno di legge su questa proposta. È già stato ricordato dai miei colleghi quanto atroce può essere per un genitore perdere un figlio per la propria colpa, per la propria disattenzione. Quindi voteremo convintamente a favore soprattutto sull'articolo 2, che contiene le disposizioni per le campagne d'informazione e di sensibilizzazione. Si tratta di un aspetto fondamentale per la prevenzione, su questo come su altri temi, a cominciare dalla salute. salute. È importante che quando succedono questi fatti atroci, non se ne parli per i soli due mesi estivi dimenticandoli nei dieci mesi successivi. Siamo completamente d'accordo anche sullo stanziamento finanziario per l'informazione.

questo suggerimento venga accolto. Purtroppo, vari emendamenti migliorativi del testo in Commissione non sono stati accolti. Ci sono stati anche dei rilievi da parte dell'Ufficio studi del Senato sugli articoli 1 e 3, ma sappiamo che in questo momento i tecnici non sono molto ascoltati. Noi comunque siamo sicuri che il Governo, al quale stiamo dando una delega in bianco, ci stupirà nel preparare nelle prossime settimane i decreti attuativi,

ho avuto la sgradevolissima sensazione di trovarmi in queste condizioni. Fino a quel giorno, consideravo sciocchi, smemorati, irresponsabili, distratti i genitori che si trovavano a morire - anche loro - nel verificarsi di quella disgrazia

"strombazzato" che in Italia, in questo momento, una coppia di ragazzi, di giovani che decidano di unirsi in matrimonio, fare il mutuo per la casa

beffa che lo sforzo che stiamo oggi compiendo in termini legislativi ricada economicamente su queste famiglie, che noi invece dobbiamo

d'Italia, attendendo il decreto attuativo di questa legge, che evidentemente sollecitiamo per una sua opportuna rapidità, è di approfittare della prossima legge di bilancio per apporre immediatamente le risorse affinché

Colleghi senatori, troppe volte di recente abbiamo letto notizie di cronaca le cui vittime erano bambini di pochi anni, lasciati - ahimè - in auto e ritrovati purtroppo dopo una giornata lavorativa

cosa può essere stato per il genitore, la mamma, il papà o l'intera famiglia: un senso di colpa che ognuno di questi genitori e familiari si porterà avanti per tutta la vita. PRESIDENTE. Senatrice Ronzulli, non dubito delle sue qualità artistiche

sottoscritto con me due emendamenti, poi trasformati in un ordine del giorno che impegna il Governo. Li ringrazio molto, così come ringrazio

Signor Presidente, colleghi senatori, apprezzo e condivido le intenzioni dei proponenti e condivido pienamente l'azione svolta in Commissione dai miei colleghi di Forza Italia. Purtroppo, l'incomprensibile blindatura del provvedimento messa in atto dalla maggioranza di Governo ha impedito modifiche a mio parere indispensabili. Condivido pienamente altresì gli ordini del giorno presentati dai colleghi Schifani, Gallone, Modena, Mallegni e De Siano, ma ritengo che delle modifiche sarebbero state necessarie.

Può apparire incredibile che qualcuno dimentichi un neonato in auto, ma, come ci viene spiegato, non si tratta solo di disattenzione o incuria. In molti casi ci troviamo dinnanzi a una vera e propria patologia quella dell'amnesia dissociativa - che si manifesta in particolari condizioni di *stress* e stanchezza. Il segnalatore acustico è un piccolo accorgimento che, come ci auguriamo tutti, consentirà di evitare eventi così drammatici, in grado di segnare per sempre la vita delle famiglie. Non bisogna mai sottovalutare i pericoli di quando si è alla guida. Dal mancato fissaggio dei seggiolini, fino all'utilizzo dei cellulari durante la guida: sappiamo tutti quanto tutto questo possa fare la differenza. Per questo motivo, sono d'accordo con la volontà del ministro Toninelli di inasprire le pene per chi viola le norme, a cominciare dal ritiro della patente per chi parla o scrive al cellulare. In Commissione si è dibattuto anche sui potenziali costi a carico dei cittadini. È importante che il Ministero, dando seguito agli ordini del giorno che la Commissione ha accolto, si adoperi per definire caratteristiche tecnico-costruttive dei sensori in un'ottica di contenimento dei suddetti costi. Perché meno costerà questo dispositivo più velocemente verrà raggiunto l'obiettivo di questo provvedimento. Ed è con questo auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

Sarà una dichiarazione brevissima, fondata su tre considerazioni. La prima: un'Assemblea che vota all'unanimità un atto di civiltà è un fatto sempre in sé positivo. La seconda delle considerazioni: assistiamo da cinque anni, dal 2013, a un fenomeno verticale di abbandono dei piccoli nelle auto. I motivi sono molti, indagati da psicologi e sociologi. Sta di fatto che questo provvedimento diventa indispensabile. È un fenomeno non soltanto italiano e infatti sono stati citati dati e numeri che riguardano gli Stati Uniti e larghissima parte anche dell'Europa. È un dato che ha a che fare con la contemporaneità e - vorrei dire - anche con una sorta di presentismo, che ogni giorno ci uccide nella valanga di grandi e piccole questioni quotidiane da cui le donne e gli uomini sono travagliati.

è stato oggetto di discussione e di riflessione nei mesi e negli anni passati e a tutt'oggi conferma, purtroppo, la sua validità: sia la mancanza di seggiolini con l'allerta per bambini sia l'uso o, anzi, la mancanza di una contravvenzione forte rispetto a chi usa lo *smartphone* o altri strumenti tecnologicamente avanzati quando si trova alla guida di una vettura stanno provocando il numero maggiore di feriti e di morti sulle strade.

i seggiolini per bambini esistenti dotandoli del meccanismo di allerta. Quell'atto, cioè la possibilità in norma di utilizzare questo meccanismo,

«Ricordo le mie urla, i miei colleghi accorrere, il loro cercare di starmi vicino e poi l'arrivo dei soccorsi, la mia disperazione senza rimedio, l'impossibilità di accettare quanto era accaduto. Il macerarmi su come fosse stato possibile. Non sono neanche riuscito a salutare mio figlio come avrei voluto. Il trauma è stato devastante». Gentile Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto iniziare il mio intervento a nome del Gruppo Fratelli d'Italia con le parole di un padre, con le parole esemplificative di un dramma che ha scosso un'intera famiglia lacerando una comunità intera, con le parole di chi ha visto scivolare via la vita del proprio figlio di due anni perché dimenticato chiuso nell'abitacolo dell'auto familiare. Ecco, la proposta di legge di cui oggi stiamo discutendo è la legge Meloni, voluta fortemente dal nostro presidente Giorgia Meloni, che saluto per la sua presenza. FdI)*. Come ricordava qualcuno, salvare un bambino è come salvare il mondo. Questo nostro impegno per la ricerca di un dispositivo che va a salvare la vita che va a salvare la vita merita la presenza di un *leader* nazionale come il nostro, che noi abbiamo la fortuna di avere qui nella nostra Aula. Ecco perché abbiamo seguito con grande attenzione il cammino di questa legge, verificandone progressivamente l'*iter*. Voglio ringraziare - come ricordava Isabella Rauti tutti coloro che non hanno creato ostruzionismo, ma che hanno voluto guardare alla *ratio* di una legge di grandissima civiltà, che pone l'Italia all'avanguardia nella sicurezza stradale e nell'importanza che va assicurata alla vita umana. Era doveroso, per noi di Fratelli d'Italia, impedire il ripetersi di queste morti assurde abbiamo voluto appunto batterci con tutte le nostre forze per la legge Meloni, perché chi dimentica - lo dobbiamo qui ricordare - spesso è vittima egli stesso di una società che pretende troppo da tutti. Non sempre dietro a questi drammi ci sono genitori negligenti, anzi quasi mai. Paradossalmente questa è una una catastrofe che tocca proprio i genitori più responsabili, quelli che lavorano, quelli che tendono a fare mille cose. Il fenomeno della distrazione genitoriale purtroppo colpisce le società moderne in una misura molto superiore a quella che le cronache riportano. Si verificano molti più casi di quelli che noi oggi siamo qui a valutare, proprio perché molti - grazie a Dio - non terminano con questo tragico finale; ma comunque accadono. Il Gruppo Fratelli d'Italia non vuole assolutamente giudicare i genitori, ci mancherebbe altro. tuttavia ricordare quello che gli analisti di tutto il mondo industrializzato vogliono sottolineare, cioè che lo *stress* di questa società moderna genera fatali *blackout* nella mente e nella psiche di tanti di noi, di tante persone. È un offuscamento temporaneo spesso devastante, troppo fatale: fretta, *stress*, affaticamento mentale, assuefazione a una realtà che spesso tendiamo addirittura non riusciamo più a contenere. I bambini vengono dimenticati nei sedili posteriori delle nostre auto perché si ritiene di averli lasciati all'asilo, si ritiene di averli lasciati a casa, si ritiene di averli lasciati a scuola. E lo sbigottimento, quello che raccontano gli analisti, a fronte e subito dopo queste tragedie, si manifesta anche nell'incredulità del genitore: il genitore sembra incredulo, il suo cervello non reagisce.

di questi agghiaccianti meccanismi mentali. In Italia abbiamo ricordato le nove vittime accertate, sette solo dal 2011: Pisa, Arezzo, Firenze, Piacenza, Perugia, Teramo. Tragedie che però si possono ripetere; drammi che richiedono la necessità di individuare delle soluzioni adeguate, la fretta di individuare soluzioni necessarie e indispensabili. Ecco perché la legge Meloni Ecco perché la legge Meloni prevede l'obbligo, per tutti gli autoveicoli su cui viaggiano bimbi, di installare sui seggiolini appropriati dispositivi che, attraverso un segnale acustico-luminoso, avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto, anche quando si spegne la macchina, così da evitare che vengano dimenticati dentro l'abitacolo. Dopo il via libera delle Commissioni trasporti di Camera e Senato, finalmente c'è questa bella giornata di politica, questa grande esperienza parlamentare che porta l'Italia a dotarsi di una legge che ci pone all'avanguardia nella prevenzione e

questo *iter* virtuoso - non leggerò i meccanismi della legge - ci consente davvero di essere oggi qui

questa è una piccola grande priorità. La legge Meloni migliorerà l'Italia e salverà la vita di un bambino, e credo che ciò sia il massimo dell'azione politica cui un Gruppo parlamentare e un intero Parlamento possano aspirare.

Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento che abbiamo condiviso con tutti gli altri Gruppi e alla cui redazione abbiamo partecipato attivamente anche con la presentazione di una proposta di legge firma della collega Caterina Bini. Siamo d'accordo con l'introduzione in Italia dell'obbligo di utilizzare un dispositivo antiabbandono sui seggiolini che trasportano i bambini in auto al nostro esame, nonostante le criticità che abbiamo già evidenziato nella Commissione trasporti e che permangono all'interno del provvedimento. D'altronde, i dati che avevamo davanti, i numeri erano impressionanti, molto preoccupanti e alcuni sono stati citati: otto casi in Italia negli ultimi anni, decine e decine negli Stati Uniti, in Israele una decina, in Francia ancora altri

che hanno evidenziato alla nostra attenzione la necessità di un provvedimento di tale natura per prevenire gli eventi tragici, *in primis* per le famiglie e poi anche per la comunità tutta. deriva la nostra adesione, la condivisione, insieme a tanti altri, di un'ottima giornata di politica e della necessità di rendere obbligatorio il dispositivo. Abbiamo condiviso tale scelta - come dicevo - e purtuttavia permangono delle criticità, delle perplessità che abbiamo manifestato e che avevamo esposto con degli emendamenti che non sono stati accolti.

Un aspetto sul quale abbiamo manifestato idee diverse e sul quale manteniamo una certa diversità di opinione è la contraddizione insita nel doppio obbligo, centoventi giorni dopo l'emanazione del decreto del Ministero dei trasporti che ne fissa le caratteristiche tecniche e comunque entro il primo di luglio. Questo doppione potrebbe creare confusione, in particolare

si recheranno presso tre ospedali a Milano, a Napoli e a Roma, regalando a cento famiglie un dispositivo antiabbandono, testimonia che questo provvedimento è condiviso e corrisponde a una necessità reale avvertita nel Paese. È chiaro che l'obbligo del seggiolino con l'allarme comporterà una spesa. E oggi gran parte del dibattito è stato focalizzato su questo aspetto. È una spesa certo più lieve - quale famiglia non spende per la tutela dei propri bambini? - ma è pur sempre una spesa.

che avevano promesso una agevolazione fino all'importo massimo di 200 euro. Così non è stato e, anzi, gli emendamenti che avevamo proposto in Commissione sono stati bocciati. Quell'agevolazione avrebbe favorito anche un altro aspetto, perché purtroppo non c'è solo il rischio di abbandono dei bambini, ma ci sono anche i bambini che, nonostante siano sui seggiolini, subiscono gravi ferite, se non altro, proprio a causa dello stesso seggiolino. Quelle risorse e quell'agevolazione avrebbero favorito anche l'acquisto di un seggiolino migliore.

In ogni caso per noi, ovviamente, non è importante il fatto che non sia stata mantenuta la promessa. Le famiglie giudicheranno e noi staremo attenti anche per il futuro.

siamo sicuri che le famiglie lo faranno anche senza l'incentivo. Per quanto ci riguarda, quindi, non focalizziamo l'attenzione, se non denunciando quello che è avvenuto, sebbene non desistiamo da questo obiettivo. Pensiamo - ma mi pare d'aver capito che non saremo gli unici - che nella prossima legge di bilancio ci possa essere un segmento di riflessione su questo aspetto, per riparare a una tale dimenticanza. Peraltro, la legge di bilancio - come é noto - interverrà prima dell'obbligo dell'allarme sui seggiolini. E lo faremo per dare alle famiglie italiane tutti gli strumenti per scegliere il miglior dispositivo che ritengono di comprare per tutelare i loro bambini. Per concludere, signor Presidente, la necessità di tutelare i più piccoli, la serenità dei genitori e il benessere della comunità sono il bene da perseguire e prevalgono sulle lacune e sulle perplessità alle quali ho fatto riferimento, che auspichiamo vengano presto risolte. Per quel bene supremo che sono i nostri figli, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del provvedimento.

tutto l'*iter,* e in particolare le audizioni alle quali il relatore ha fatto riferimento, e hanno avuto la responsabilità e la sensibilità di

che un ritardo ulteriore nell'approvazione del testo potrebbe comportare. Spesso, sia fra gli addetti ai lavori sia nell'immaginario collettivo, le leggi vengono divise tra leggi importanti e leggi minori. Cos'è che misura, però, l'importanza di un atto? Non credo siano i fondi stanziati o il clamore suscitato. Credo che l'importanza di un atto sia data dalla capacità di leggere il proprio tempo e di dare risposte ai problemi del proprio tempo e il disegno di legge in esame risponde a tutte e due queste caratteristiche. Mi permetto di esprimere un giudizio così netto, perché uno di quei bambini, che il senatore Santillo ha ricordato per nome in Assemblea, lo conoscevo, perché era del mio paese paese e andava all'asilo con mio figlio. Conoscevo lui, conoscevo i suoi genitori

che l'importante è quanto stabiliamo all'articolo 2 nell'individuare dei fondi per la campagna di sensibilizzazione, perché - permettetemi la sanzione più grande non è la multa: la sanzione più grande che può capitare a qualcuno che vive un'esperienza del genere è dover convivere, non tanto e non solo con la morte del proprio figlio, ma col sentirsi responsabile di quella morte

un'ultima considerazione. Quest'atto è fondamentale, ma la vera risposta a un problema come quello in esame non sarà data dalla presenza in ogni auto di un dispositivo antiabbandono, avrà quando questo Parlamento sarà in grado di far sì che nella nostra società, nella nostra comunità, un papà e una mamma non siano lasciati soli, non si trovino nella condizione di scordarsi del proprio figlio *(Applausi di avere il dispositivo che glielo ricorda, ma di vivere in una società che dia risposte e sia veramente a misura di bambino, di famiglia, di papà

a vigilare perché il decreto attuativo sia emanato perché si trovino fondi ulteriori. Sappiamo benissimo che quelli stanziati servono ad aprire il capitolo per le campagne e dedichiamo questo voto - siamo convinti sarà un anime - a tutti quei genitori che, di fronte al lutto che li ha colpiti, hanno scelto non di chiudersi in se stessi, ma di chiedere per anni una legge per gli altri, perché oramai la tragedia l'avevano vissuta; e hanno chiesto

Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole, ma sarà un sì di responsabilità e non totalmente convinto, per i motivi che ora

alla Camera nella precedente legislatura la collega Giammanco da deputata aveva ottenuto l'approvazione da parte di quel ramo del Parlamento di un importante disegno di legge sull'obbligo della videosorveglianza negli asili, proprio per concentrare l'attenzione su quelle deturpazioni della dignità dei minori che sfuggivano al controllo dell'opinione pubblica e dei vigilanti. Ci stanno a cuore i minori, ma ci sta a cuore anche quella società la quale da domani, quando il provvedimento entrerà in vigore, si vedrà imposto un onere; un onere etico, un onere condivisibile sotto il profilo sociale della dignità e della serenità del minore, ma un onere anche di carattere economico.

perché si focalizzasse una particolare attenzione al criterio della economicità dei nuovi costi che si imponevano alle famiglie. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito. Abbiamo ottenuto una chiusura da parte di un Governo che ha blindato un testo - ricordiamocelo - di iniziativa parlamentare e non governativa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Questo è un fatto - secondo me - signor Presidente, anche riprovevole e grave sotto il profilo della nostra storia parlamentare. La sua storia ci ricorda quanto lei, essendo stato Ministro, conosca - come il sottoscritto, e come tanti di quelle che sono le regole non scritte ma che fanno parte del buon funzionamento delle istituzioni. Un disegno di legge di iniziativa parlamentare va rispettato perché nasce dall'iniziativa del Parlamento e non può un Governo blindare un testo dicendo che non si approva alcuna modifica. un fatto senza precedenti rispetto a modifiche di buonsenso, signor Sottosegretario, che noi chiedevamo. Bene: non le abbiamo ottenute. Abbiamo, per fortuna, ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo - senza la famosa frase critica: «invita il Governo a valutare» - a indirizzare questo testo a criteri di economicità, perché ci sta a cuore anche la serenità delle famiglie sotto il profilo di carattere economico. ci preoccupa di questa vicenda? Ci preoccupa l'approccio dell'Esecutivo su questo tema, e non vorremmo - lo diciamo sin da adesso - che questa modalità si potesse ripetere. Vede, signor Presidente, questo Governo, dinanzi ai grandi problemi che si sono verificati negli ultimi mesi - mi riferisco alla tragedia del crollo del ponte di Genova, come ad altri temi - anziché rassicurare il Paese e individuare le soluzioni, ha individuato un nemico da abbattere, sul quale ha scaricato le tensioni e la possibilità delle soluzioni.

una riflessione sulla rimozione immediata, da parte del Governo, della direttrice del carcere di Rebibbia all'indomani di un evento che ci ha sconvolto: una detenuta nigeriana uccide i propri figli per disperazione. Non entro nel merito del reato, ma mi sarei aspettato dal Governo non tanto la sospensione,

Mi sarei aspettato anche una parola più rassicurante da parte del presidente del Consiglio Conte quando il suo portavoce - lo sappiamo tutti - ha indotto un collega ad

Dico soltanto, signor Presidente, che, se Paolo Bonaiuti, portavoce di Silvio Berlusconi, avesse proferito quelle espressioni, si sarebbe scatenato il finimondo, non tanto nei confronti di Paolo Bonaiuti ma nei confronti del presidente dell'epoca Silvio Berlusconi. *(Commenti dal Concludo dicendo che stigmatizziamo il comportamento del Governo su questo argomento che ci sta a cuore e voteremo favorevolmente, ma ci faremo sentire con le nostre iniziative legislative. Porteremo in Assemblea le nostre proposte e verificheremo se vi è la volontà di questo Governo, o da parte di alcune forze di Governo, di condividere le nostre proposte di centro-destra.

sottosegretario Dell'Orco, onorevoli colleghi, prima di affrontare questo importantissimo provvedimento, vorrei raccontarvi una breve storia: quella di Gaia e del suo papà. Francesco era un ottimo avvocato, ma soprattutto il padre migliore del mondo, molto attaccato alla famiglia e alla figlioletta Gaia, Nell'agosto di qualche anno fa, Francesco stava vivendo un durissimo periodo lavorativo con conseguente forte *stress*. Un venerdì mattina, dopo l'ennesima nottata passata senza dormire, salutò la moglie, prese la bimba in braccio e decise di portarla lui al nido. seggiolino nel sedile posteriore e si avviò. Faceva un caldo insopportabile. Francesco arrivò trafelato e parcheggiò l'auto in un ampio spazio distante dalla via principale. Prese la valigetta riposta sul sedile anteriore e corse verso il suo ufficio. La piccola Gaia, dunque, rimase lì dentro, sotto quelle lamiere che nel giro di cinque minuti iniziarono ad assorbire i raggi solari, facendo diventare l'auto un forno crematorio. In quel momento Gaia si svegliò rossa in faccia e tutta sudata. I bambini a quest'età non capiscono molto, ma hanno una vaga idea della sensazione di pericolo. Gaia iniziò a cercare con lo sguardo il suo papà. Le sue orecchie sentivano solo vuoto e silenzio. Iniziò a piangere, a lamentarsi di quel caldo insopportabile, per quell'esperienza che mai avrebbe voluto vivere. Si sentiva sola, abbandonata, in pericolo. Dopo quindici minuti all'interno dell'auto il caldo divenne asfissiante, intorno ai 50 gradi. Lei era intrappolata, incollata con la schiena al seggiolino che la immobilizzava col volto verso il sole che si faceva sempre più forte; il suo pianto era incessante, la sua temperatura corporea saliva sempre di Affannava, aveva fame d'aria, il respiro era accelerato. Poi a un certo punto smise pure di piangere, perché non ci riusciva più. Gaia si stava addormentando per l'ultima volta, mangiata dal sole, in un'auto incandescente. Dopo sette ore Gaia non respirava più, non pensava più. Dopo sette ore Gaia era morta. Dopo otto ore il papà uscì dal lavoro, aprì l'auto, fece per mettere dietro la valigetta allorquando vide la scena che un papà non vorrebbe mai vedere. Svenne e si risvegliò in ospedale, circondato da infermieri e poliziotti, con una notifica per omicidio colposo. La sua vita era finita per sempre. Francesco, infatti, non si è mai più ripreso. Onorevoli colleghi, mentre scrivevo il discorso non nascondo che i miei occhi sono diventati lucidi più volte. Ho pensato a quella creatura di Dio, a quanto possa aver sofferto. E ho pensato anche ai genitori, ma soprattutto al papà. Quel giorno è morta non soltanto Gaia, ma un intero nucleo familiare. Negli ultimi anni in Italia non sono morti solo una decina di bambini. Negli ultimi anni in Italia sono morti una decina di bambini più le loro famiglie. Negli ultimi sedici anni, sono morti per questa causa oltre 620 bimbi. Solo negli Stati Uniti ogni dieci giorni un bambino dimenticato in auto in auto muore a causa di un colpo di calore. Sapete cosa ha fatto il Governo statunitense? Ha realizzato e trasmesso degli *spot* toccanti e di forte impatto, che mostrano tutte le fasi della tragedia, le stesse fasi che ho voluto raccontarvi qui oggi in Senato. Parliamo di tragedie derivanti per lo più da fatali distrazioni attribuibili allo *stress*, a ritmi insostenibili di lavoro, ad una vita quotidiana sempre più asfissiante e dominata da una società che sta schiacciando le vite di famiglie normali. Eppure, parliamo di tragedie facilmente evitabili, grazie alla semplice introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per evitare l'abbandono dei bambini nelle auto. A tal proposito, c'è stata una proposta di legge nel 2014, nonché un disegno di legge già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. deputati. L'articolo 172 del nuovo codice della strada prevede che i bambini di statura inferiore al metro e mezzo devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta. Col disegno di legge su cui siamo chiamati a esprimerci, si interviene proprio su questo articolo, prevedendo l'obbligo per tali sistemi di ritenuta, al fine di essere equipaggiati con un dispositivo di allarme antiabbandono. Parliamo di tecnologie atte a rilevare e a segnalare acusticamente la presenza di bimbi seduti nei seggiolini allorquando si chiude la portiera dell'auto. La Camera dei deputati ha già approvato all'umanità il disegno di legge n. 766. All'articolo 3 il disegno di legge prevede che l'acquisto di questi dispositivi possa essere facilitato da agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, in ossequio a una disciplina successiva che fisserà in concreto le suddette agevolazioni. Ovviamente queste tecnologie saranno poi rese obbligatorie nei seggiolini in vendita, così da sgravare i conducenti dell'onere connesso all'adempimento del disegno Inoltre, l'approvazione oggi del provvedimento in Senato permetterebbe di rispettare la scadenza del 1° luglio 2019 prevista per la piena efficacia dell'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme, in virtù del decreto ministeriale contemplato proprio dal disegno di legge n. Certe battaglie non hanno colore politico; certe battaglie devono essere d'esempio per la collettività. Io guardo Gaia e penso a mia figlia. Sono una persona normale, spesso stressata proprio come papà Francesco. Quella tragedia avrebbe potuto cogliere anche me, così come ognuno di voi. Siamo fallaci, siamo deboli. Possiamo commettere errori perché siamo umani. Io credo che il sorriso di un bambino possa valere il costo di un dispositivo salvavita. Credo che poter vedere mia figlia crescere, sposarsi e partorire i miei nipoti possa valere il costo di 100 euro a IVA agevolata. Occasioni come quella di quest'oggi ci devono vedere tutti uniti, al di là del colore politico; ci devono vedere Stato, istituzioni anzitutto e, soprattutto, genitori responsabili. Dichiaro, signor Presidente, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento in oggetto. Il mio invito è a votare non solo con la testa, ma soprattutto con il cuore che

Vi rendete conto della responsabilità che ci stiamo per assumere? Vi rendete conto che Gaia avrebbe potuto essere vostra figlia? Onorevoli colleghi, oggi potrete decidere se impedire la morte della prossima Gaia o esserne corresponsabili.

alla 5a Commissione permanente di concludere l'esame in sede referente dei disegni di legge di rendiconto 2017 e assestamento 2018. Il termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea per i predetti provvedimenti è fissato per le ore 10 di domani. Comunico inoltre che domani, alle ore 9,30, avrà luogo una riunione del Presidente del Senato con i Presidenti delle Commissioni permanenti e che alle ore 12 è convocata la Conferenza dei Capigruppo.

al Sud delle Marche, all'Abruzzo, al Molise e al Nord della Puglia. Poiché c'è una scadenza (entro il 31 dicembre di quest'anno), occorre concludere l'attività istruttoria ad opera dello Stato membro, cioè dell'Italia, nei confronti della Commissione.

Signor Presidente, svolgo il mio intervento anche a nome delle colleghe Nisini e Sbrana per segnalare quello che sta succedendo oggi a Pisa: